credo molto nel telelavoro e nell'aiuto che l'innovazione tecnologica può dare all'inclusione delle donne all'interno del mercato del lavoro, ed in particolare alle donne con disabilità. Per facilitare soprattutto l'accesso delle donne con disabilità al mercato del lavoro si potrebbe privilegiare la destinazione delle risorse ad iniziative che considerino queste donne come utenti prioritari. La disabilità è un tema al quale prestiamo particolare attenzione; nei giorni scorsi è stata avviata una campagna di comunicazione dal titolo: «Abilità diverse, stessa voglia di vita», per contrastare il fenomeno dell'esclusione e della discriminazione nei confronti dei disabili. Si tratta di una campagna che racconta con un linguaggio molto semplice, un linguaggio simbolico, una verità di cui a volte ci dimentichiamo: una disabilità può impedire ad una persona di fare qualcosa, non può impedire ad una persona di fare tutto. Sarà ovviamente cura del Dipartimento per le pari opportunità, anche attraverso ulteriori campagne informative, garantire la promozione unitaria delle linee di intervento più innovative che meritano maggior impegno di divulgazione e di sensibilizzazione. È stato poi avviato con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione e il Sottosegretario per le politiche della famiglia un progetto pilota di apertura di nidi aziendali presso le sedi centrali e periferiche delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di favorire l'incremento del numero dei nidi di infanzia e dei posti nidi d'infanzia esistenti sul territorio nazionale, nonché di promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno alle famiglie, distribuendo così i carichi di cura e favorendo la parità tra uomini e donne e contestualmente favorendo la flessibilità nel mercato del lavoro. Anche nel piano "Italia 2020" per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro, che abbiamo elaborato d'intesa con il ministro Maurizio Sacconi, sono previste cinque linee di azione che hanno come obiettivo quello di favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. Se poi spostiamo l'attenzione all'impianto normativo e di tutela della madre lavoratrice nel confronto internazionale e comparato, l'Italia senza dubbio presenta una delle legislazioni più avanzate del mondo e pienamente in linea con la normativa comunitaria. Basti pensare che a livello europeo si sta discutendo oggi di una direttiva rispetto alla quale l'Italia è già assolutamente in linea. Riconosco tuttavia che le lavoratrici dipendenti godono di un regime più favorevole rispetto alle donne imprenditrici, e quindi condivido la proposta di legge della senatrice Laura Bianconi, volta a consentire alle lavoratrici autonome, nel periodo di astensione per maternità, la contribuzione di tipo parzialmente figurativo. La questione peraltro riguarda non solo le imprenditrici, ma anche le libere professioniste. gennaio 2010, n. 5, di recente varato per il recepimento della direttiva 2006/54/CE, relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, prevede tra l'altro il divieto di discriminazione per ragioni connesse al sesso, allo stato di gravidanza, di maternità o di paternità, anche adottive. Si interviene inoltre sul cosiddetto *gender pay gap*, vietando qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, relativa alle retribuzioni, sanzionando i datori di lavoro che discriminano le lavoratrici con l'ammenda da 250 a 1.500 euro e stabilendo altresì, qualora il datore di lavoro non ottemperi alla sentenza che accerta la discriminazione, l'ammenda fino a 50.000 euro e l'arresto fino a sei mesi. sottolineare, e mi avvio alle conclusioni, l'impegno del Governo per il rilancio di misure di sostegno all'imprenditoria femminile, specialmente nel Mezzogiorno. La legge n. 215 del 1992 è ora in una fase di stallo, non per volontà del Governo Berlusconi, ma perché non è stata rifinanziata da parte di molti Governi. Il limite dell'attuazione di quella legge - bisogna dirlo - è stato tuttavia quello di concedere finanziamenti a pioggia, senza una seria regia e senza un monitoraggio costante degli effetti in termini di incremento dell'occupazione femminile. La mia idea, la nostra idea, alla quale stiamo lavorando con il Ministro dello sviluppo economico nel quadro più ampio del piano del Governo per il Sud, è quella di reperire nuove risorse ricorrendo a fondi europei per favorire l'accesso al credito delle imprese femminili operanti nel Mezzogiorno attraverso l'utilizzazione della garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese, di cui alla legge n. 662 del 1996, ed un contributo non più in conto capitale ma in conto interessi. Il nostro impegno anche in questa direzione è forte e costante, ma più in generale l'impegno del Governo Berlusconi per per favorire l'inclusione delle donne all'interno del mercato del lavoro è un impegno che, come ho affermato in apertura, oserei definire prioritario.

per favorire l'occupazione femminile e il potenziamento dei servizi per la prima infanzia su tutto il territorio nazionale. Ad oggi, però, purtroppo, provvedimenti attuativi non ci sono stati in tal senso, tanto che nella Commissione lavoro del Senato sono stati presentati sull'argomento ben tre disegni di legge da parte dell'opposizione, ai quali ultimamente se ne è aggiunto uno della maggioranza. Tali proposte sono state molto apprezzate e condivise in sede di audizione dalle parti sociali e da diverse associazioni femminili. Ci auguriamo che lei con il suo Governo dia un chiaro

Signora Presidente, signora Ministro, sappiamo bene che la scarsa presenza delle donne nelle istituzioni e nei luoghi decisionali non si può considerare come un mero problema di settore relativo al cattivo funzionamento della politica, superabile attraverso una serie di aggiustamenti tecnico-giuridici. Questa condizione altamente discriminante per le donne si ripercuote visibilmente nella scarsa attenzione alle pari opportunità da parte delle istituzioni che non riescono a vedere le diverse necessità, e quindi a rispondere alle differenti esigenze della donna cittadina rispetto a quelle dell'uomo cittadino. A questo proposito le chiedo, onorevole Ministro, quali provvedimenti il Governo intenda porre in essere per garantire che in tutti i settori in cui si prendono decisioni, in primo luogo nelle istituzioni, venga rispettata la giusta rappresentanza delle donne, che continuano ad essere in proporzione ancora troppo poco rappresentate. Ne ha facoltà. CARLONI *(PD)*. Signora Presidente, onorevole Ministro, le recenti elezioni regionali hanno visto confermato un triste primato italiano: quello della bassa presenza di donne nelle assemblee elettive. A parole tutte e tutti si dichiarano concordi sulla necessità di colmare il grande divario che esiste tra società civile ed istituzioni della politica, tra presenza maggioritaria delle donne nel corpo elettorale e nella vita socio-culturale a fronte del mancato riconoscimento nelle assemblee elettive. Nei fatti in Italia non si è ancora data attuazione al principio sancito dall'articolo 51 della Costituzione in materia di promozione di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive. Bisogna tornare al 2005 per ricordare l'ultima volta in cui, a lungo e inutilmente, si è posta in Parlamento la questione di prevedere un meccanismo che garantisse una presenza femminile nella legge elettorale nazionale per il rinnovo del Parlamento: il risultato è stata una legge elettorale che in nessun modo consente agli elettori di pronunciarsi sulle candidature, né favorisce la presenza delle donne nelle liste. L'unica eccezione è rappresentata si è dotata di una legge elettorale che, con un rimedio semplice ed ineccepibile sotto il profilo costituzionale (quello della doppia preferenza uomo-donna), ha dato buoni frutti, consentendo l'elezione di 14 donne su 60 in Consiglio regionale. Alla luce di questa positiva esperienza, ritiene di doversi impegnare per cambiare le leggi elettorali nazionali, provvedimento che, tra l'altro, non avrebbe oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato?

disquisire con noi su un tema così importante come quello della rappresentanza delle donne nelle istituzioni. Come il Ministro sicuramente saprà, è stato recentemente

nelle istituzioni come elemento per garantire la stabilità e la crescita economica dell'Europa. In questo rapporto, però, la Commissione europea ritiene che le donne siano scarsamente rappresentate nelle posizioni *senior* delle istituzioni.

nelle posizioni decisionali della politica, della finanza e delle istituzioni in generale. La rappresentanza femminile nelle ultime elezioni del Parlamento europeo è stata molto importante, ma non vi è un riscontro altrettanto importante nelle istituzioni dei singoli Paesi, in primo luogo nel nostro Paese,

la rappresentanza femminile sia più importante non solo dal punto di vista numerico, ma anche qualitativo, cioè affinché le donne possano accedere a quelle posizioni *senior* in cui oggi sono sottorappresentate. [POLI

D'altra parte, anche quando c'è stata l'opportunità di quella legge - che non condividiamo assolutamente - per la quale noi qui dentro siamo nominati,

date dalle norme, non si vuole intervenire per rendere più efficace la presenza femminile all'interno delle istituzioni.

Che ricetta ha lei, Ministro, per fare in modo che le donne, dopo tanti anni

Onorevoli senatrici e senatori, permettetemi innanzitutto di richiamare in apertura quanto affermato dal presidente del Senato, l'onorevole senatore Schifani, nel corso del recente convegno organizzato dalla Commissione per la parità e le pari opportunità di Palazzo Madama. Non sono solo le donne ad avvertire l'esigenza di essere maggiormente presenti ed attive nei circuiti dirigenziali, ma è la società intera ad avere fortemente bisogno di una maggiore presenza femminile affinché venga raggiunto quell'equilibrio necessario alla costruzione di un modello europeo di democrazia matura. Il dibattito relativo alla partecipazione delle donne nelle istituzioni sicuramente è molto attuale; investe la questione della democrazia paritaria e non c'è dubbio che occorre dare efficace attuazione anche nelle istituzioni politiche all'articolo 51 della Costituzione che garantisce il diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e prevede che la Repubblica promuova con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne. Bisogna dire che esiste finalmente oggi quello che è stato definito un vero e proprio statuto delle pari opportunità, che si articola in norme internazionali (come per esempio la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna), norme comunitarie (da quelle contenute all'articolo 23 della Carta di Nizza al Trattato di Lisbona), norme nazionali (dagli articoli 3 e, soprattutto, 51 della Costituzione al codice delle pari opportunità), che hanno come obiettivo quello di raggiungere la parità uomo-donna in tutte le cariche pubbliche, comprese quelle elettive. Tuttavia, bisogna ammettere che, nonostante il riconoscimento formale dei diritti politici, le donne non sono ancora riuscite ad entrare a far parte in misura consistente delle istituzioni politiche rappresentative. Si tratta di un fenomeno trasversale - occorre dirlo - che coinvolge tutti i Paesi del mondo indistintamente, a dimostrazione del fatto che ancora forse nessuno ha trovato quella ricetta miracolosa che possa garantire ed affermare un principio sacrosanto di equità e di giustizia sociale. In media, nei Paesi dell'Unione europea, la partecipazione politica femminile è piuttosto bassa, fatta eccezione per i Paesi scandinavi in cui, grazie a delle precise azioni positive, si è riusciti a raggiungere un alto tasso di presenza delle donne nelle sedi ufficiali della politica ed in professioni di alto impegno, al punto da far ritenere in Svezia le rigorose legge ivi approvate a partire dal 2003 ormai superate, addirittura dannose per le donne stesse. Nel Parlamento europeo, la presenza femminile si attesta intorno al 40 per cento, che è un dato decisamente al di sotto della componente femminile della popolazione, anche se è più che raddoppiata rispetto agli anni Ottanta. La media della componente femminile nei Governi nazionali è invece pari al 24 poco al di sopra delle percentuali di Ministri donne nel Governo italiano, e scende dal 21 al 16 per cento se si considerano anche Vice Ministri e Sottosegretari. I motivi della scarsa presenza delle donne nelle istituzioni rappresentative sono diversi, legati sia alla crisi della rappresentanza, sia a fattori socio-culturali, che richiedono una forte sensibilizzazione dell'opinione pubblica ed una modifica della cultura politica, che ancora oggi considera l'uomo come il solo legittimo protagonista della gestione dello Stato. Ritengo quindi che la presenza delle donne nelle istituzioni sia un obiettivo necessario ed utile all'intera collettività. In Italia, le donne sono oltre la metà degli aventi diritto al voto, ma non sono mai riuscite a superare la quota di un quarto delle persone elette. Nel corso degli anni, la percentuale delle elette al Parlamento non ha avuto un andamento lineare, rimanendo comunque nella media del 7-9 per cento, fino all'XI legislatura, e salendo alla quota del 15 per cento nel corso della XII legislatura. Ed è solo dopo il 2003, con la modifica dell'articolo 51 della Costituzione, che la rappresentanza delle donne in Parlamento riprende pian piano a crescere. Dai dati aggiornati al 16 aprile 2010, risulta che in Parlamento ci sono 193 donne: 59 senatrici e 134 deputate; tra queste, 62 appartengono alla maggioranza e 60 al Partito Democratico, quattro all'UDC, due all'Italia dei Valori e due al Gruppo Misto.

Anche se il *trend* è indubbiamente positivo, a livello internazionale questi dati posizionano il nostro Paese solo al cinquantaduesimo posto su 188 Nazioni, al pari della Cina e dietro Paesi come Argentina, Cuba, Spagna, Germania, Nuova Zelanda, Svizzera e Portogallo. Queste percentuali di rappresentanza femminile sono lontane rispetto alla soglia del 30 per cento stabilita dalla Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile già nel 1990 e considerata come quota minima affinché le donne possano realmente avere un peso decisionale. Se poi spostiamo l'attenzione a livello regionale, nel 2009 la presenza femminile nelle Giunte e nei Consigli regionali superava di poco il 12 per cento. In base ai dati delle ultime elezioni regionali, le consigliere elette sono il 13,3 su 697 eletti nelle 13 Regioni andate al voto, 93 sono donne. Nel Lazio, le consigliere regionali sono 12; in Piemonte, su 50 eletti, ci sono 14 donne: 8 del centrodestra e sei del centrosinistra; in Campania, su 61 consiglieri, 14 sono donne: 10 del centrodestra e 4 del centrosinistra. Anche se l'andamento, pur lento, è costantemente in direzione favorevole alla partecipazione femminile, siamo senza dubbio ancora molto, troppo lontani dall'obiettivo del 30 nonostante alcune leggi elettorali regionali abbiano mostrato attenzione per la questione della democrazia paritaria, riservando al genere sottorappresentato una percentuale di posti in lista (dalle misure più blande della Calabria, che prevedono la misura minima di non discriminazione, a quelle della Puglia, del Lazio, delle Marche, della Toscana e dell'Umbria, che prevedono la riserva di un terzo), o prevedendo, come la Regione Campania, che le due preferenze vadano obbligatoriamente destinate a rappresentanti di due generi, a pena di annullamento della seconda preferenza. sottolineare che la partecipazione politica non è verificabile solo attraverso un'analisi quantitativa dei dati, bensì è un fenomeno multidimensionale, che si esprime a diversi livelli di partecipazione, istituzionalizzata e non, visibile e non. Spesso, infatti, l'interesse verso il mondo politico e la cosa pubblica non necessariamente si traduce in attività di sostegno alla politica in senso stretto o in un'attività con chiara visibilità all'esterno. (denominata «Aspetti della vita quotidiana»), realizzata dall'ISTAT dall'8 marzo 2010 e riferita all'anno 2009, è stata analizzata la cosiddetta partecipazione politica multidimensionale delle donne. Negli ultimi dieci anni, secondo i dati ISTAT, le donne che parlano di politica almeno una volta alla settimana sono cresciute del 46,9 per cento, più del doppio degli uomini; quelle che si informano di politica almeno una volta alla settimana sono cresciute del 20 per cento; quelle che si informano tutti i giorni del 25 per cento; cala il numero di persone che non ne parla mai e, anche in questo caso, soprattutto tra le donne. Nella consapevolezza di quanto sia importante avvicinare le cittadine alle istituzioni pubbliche e politiche, il Dipartimento per le pari opportunità, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la collaborazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ha promosso la realizzazione di un percorso formativo denominato «Donne, politica e Grazie L'iniziativa è stata finanziata dal Dipartimento e dagli atenei al 50 per cento; sono state 35 le università che hanno aderito e circa 2.800 i frequentatori, uomini e donne, dei corsi di formazione. L'obiettivo del progetto è stato quello di fornire un insieme di conoscenze, in parte teoriche, in parte pratiche, per diffondere la cultura di genere. Inoltre, il progetto ha voluto promuovere l'affermazione e la partecipazione nella vita politica e sociale delle donne, che rappresentano un patrimonio prezioso di risorse umane nel nostro Paese. L'offerta formativa ha insistito sulle conoscenze attinenti al funzionamento di determinati meccanismi istituzionali, politici e di *governance* ed è allo studio una nuova edizione di questo progetto. Anche nella pubblica amministrazione, nonostante la componente femminile sfiori il 50 per cento del totale, le dirigenti di seconda fascia si fermano ad un 25 per cento ed i dirigenti di prima fascia restano ancora più indietro. A livello di amministrazione centrale, la presenza delle donne nelle posizioni dirigenziali è un po' più alta. Le dirigenti generali di seconda fascia sono il 35 per cento, le dirigenti di prima fascia sono il 20 per cento. Per assecondare un percorso di crescita delle donne anche nelle posizioni apicali della pubblica amministrazione, ho chiesto e ottenuto dal ministro Brunetta che uno degli indici di valutazione delle *performance* delle amministrazioni fosse proprio la promozione delle pari opportunità. Anche instaurando un meccanismo premiale, infatti, credo si possa incoraggiare un circolo virtuoso a vantaggio di una maggiore presenza femminile nei processi decisionali. intraprendere? Come fare a garantire una maggiore presenza delle donne all'interno delle istituzioni e del mondo politico più in generale? Personalmente sono d'accordo con la senatrice Poli Bortone: non credo alle quote rosa, preferisco che la scelta ricada sulle donne per i loro meriti. Non possiamo certo credere che manchino talenti femminili se è vero, come è vero, che nel 2009 ben cinque premi Nobel sono stati assegnati alle donne. tuttavia di affermare - credo che questo sia il compito più difficile che ci spetta - una nuova cultura che prenda coscienza dei valori, dei talenti e dell'indispensabilità del contributo che le donne possono portare nei processi decisionali. Si deve puntare su azioni positive strategiche e su azioni di sensibilizzazione. Le prime devono essere rivolte a ottenere un risultato effettivo, misurabile, duraturo, strutturale e di sistema; le seconde devono prevedere interventi nella formazione anche politica e nell'informazione, per diffondere la promozione della figura e del ruolo femminile nel tessuto delle istituzioni, in modo da garantire una presenza equilibrata a tutti i livelli decisionali e in tutti i settori. Un'informazione non solo per le donne ma anche alle donne, perché divengano sempre più consapevoli del ruolo fondamentale

che abbiamo incontrato le dipendenti CAI. Stiamo cercando, tra mille difficoltà, di ottenere l'esonero dal lavoro notturno per le madri lavoratrici. Inoltre, accolgo con favore l'idea di istituire un organismo di vigilanza cui le donne possano rivolgersi per segnalare eventuali discriminazioni che fossero costrette a subire. PRESIDENTE. Hanno

che se, da una parte, come lei stessa ha sottolineato, sono ancora ben lontani dagli obiettivi stabiliti, registrano comunque un nuovo incremento della rappresentanza femminile nelle istituzioni.

Auspico che si affermi quella cultura delle pari opportunità - come lei ha detto, signora Ministro - che si fonda sui principi della nostra Carta costituzionale, ma auspico anche da parte sua un'attenzione per i disegni di legge

onorevole Ministro, la ringrazio per la sua risposta anche se, per la verità, ritengo che lei abbia scelto in questa sede di non rispondere alla domanda che le ho formulato, ovvero se lei intende impegnarsi per modificare le leggi elettorali nazionali. Auspico comunque che lei voglia pensare a questo, considerando appunto il buon esito delle recenti elezioni in Campania, dove è stata possibile l'elezione di tante donne, pur senza pensare a meccanismi di quote, e considerando che l'anno prossimo voteranno importanti amministrazioni locali e che in molti casi esistono Comuni dove non c'è una donna eletta. Quindi la invito a riflettere e a considerare anche da questo punto di vista le iniziative legislative presentate nell'attuale legislatura. Tra l'altro, la invito a considerare l'opportunità di proseguire sulla strada di promozione della cultura delle pari opportunità, anche confermando i comitati di pari opportunità nella pubblica amministrazione, rispetto ai quali mi sembra che il Governo, invece, stia procedendo a scelte diverse.

Rilevo però che, rispetto alla situazione estremamente critica che lei ci ha rappresentato, l'azione del Governo fino ad oggi svolta, che dalle sue parole apprendo essere limitata a momenti formativi, sia assolutamente insufficiente rispetto agli obiettivi che credo tutti ci poniamo. La invito, ma in modo un po' più forte rispetto a come hanno fatto le mie colleghe, ad analizzare e a far visionare dai suoi uffici tutte le proposte di legge che giacciono da diverse legislature, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica, che potrebbero essere un punto di avvio anche di azioni azioni successive da parte del Governo. Si tratta di disegni di legge che vengono riproposti ad ogni legislatura e che non trovano mai uno sbocco concreto. Quindi, come impegno concreto, signora Ministro, le chiedo veramente di fare questo lavoro di analisi di analisi delle proposte esistenti, perché da lì possiamo partire in modo serio e concreto. Ministro, la ringrazio, anche a nome della collega Bianchi, per l'attenzione che ha voluto riservare alle nostre indicazioni ed anche per aver ricevuto le lavoratrici di Alitalia. Sappiamo che dovrà fare una bella fatica, anche perché ci sono i sindacati, che non mi sembra siano particolarmente vicini a queste tematiche. Siamo qui anche per dirle che presteremo grande attenzione a tutto ciò che riguarderà quello che lei ha voluto riferire in quest'Aula: l'attenzione del Governo ai temi della formazione ed anche alla creazione di una nuova cultura e di una forte sensibilizzazione nei riguardi di quella che può essere realmente una cultura delle pari opportunità. Quindi, senza pregiudizio alcuno, affronteremo qualunque tipo di iniziativa questo Governo vorrà offrire all'attenzione dell'Aula, con l'auspicio che si possa anche convergere rispetto ad alcune tematiche che, a quanto registriamo, stanno a cuore a tutti noi.

Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della giustizia:* «Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania»